Essa presenta alcune condivisibili innovazioni, ma anche elementi di grave criticità che spesso mettono in discussione le migliori intuizioni riformatrici che il testo intendeva sottolineare. È pur vero che questa riforma viene varata nel bel mezzo di una crisi straordinaria che, oltre che economica e finanziaria, è soprattutto culturale. Siamo e saremo sempre più costretti a ridisegnare il modello della società occidentale in cui siamo inseriti, modificando il nostro stile di vita e, soprattutto, razionalizzando in ogni settore della società, puntando su ciò che serve veramente e ciò che veramente vale sia per l'interesse individuale, che per quello collettivo. Il cambiamento che la crisi ci chiede impegna in particolare il mondo universitario a cimentarsi su una proiezione di tipo internazionale su cui presenta un grave deficit, basata sulla cultura del merito, non tanto declamata quanto realmente applicata e soprattutto economicamente sostenuta. Il testo, che ad una prima lettura può sembrare coraggioso, è invece per alcuni aspetti conservatore e centralistico. Abbiamo già visto, purtroppo, altre riforme (cito, fra tutte, quelle della Moratti e quella di Berlinguer) entrare in Parlamento con un forte carico di novità ed uscirne completamente ridisegnate e sfigurate da presunte o pesanti zavorre conservatrici e corporative. La nostra università è la sede privilegiata per la ricerca e lo sviluppo culturale del nostro Paese. Essa non può che essere l'asse strategico della politica di un governo intelligente, che decidendo di puntare sullo sviluppo e la competitività internazionale non può che finanziare adeguatamente il sistema universitario, modificandone i meccanismi di *governance* e di reclutamento per valorizzare le migliori energie dentro la cornice di una autonomia fondata sulla responsabilità. Così invece non è. Rispetto alle esigenze del cambiamento, la riforma non è supportata da adeguati finanziamenti. Facciamo rilevare che, oltre ai pesanti tagli che incidono fortemente sulla qualità del sistema universitario e in particolare nella didattica e nella ricerca, che non sono più tollerabili, i 2,5 milioni che vengono investiti per la chiamata diretta nei ruoli della docenza di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero (a fronte di un miliardo di euro che ogni anno vengono sprecati rispetto alla voce più importante, che è il capitale umano: parlo dei cervelli in fuga che forniamo ma non riusciamo a recuperare dagli altri Paesi), sono una goccia che che si perde nel mare della necessità e dell'urgenza di scelte che ancora una volta non si ha il coraggio di compiere fino in fondo. abbiamo continuamente perso terreno poiché le nostre università non sono riuscite a stare al passo con gli obiettivi di Lisbona, sia per la mancanza di una seria riforma ordinamentale, che per mancanza di finanziamenti adeguati. Siamo tra gli ultimi Paesi d'Europa per la spesa in formazione e ricerca (lo 0,8 per cento del PIL grida vendetta rispetto agli altri Paesi europei). La riforma 3+2 (targata Berlinguer-Zecchino) è stata criticata e bocciata dalla nostra magistratura contabile sia per il dispendio delle risorse, sia perché non ha prodotto aumento di laureati, né il miglioramento dell'offerta formativa; essa è servita solo all'inutile e dannoso proliferare delle cattedre e a dequalificare il percorso formativo, poiché quasi tutti gli studenti hanno proseguito negli studi. L'università deve tornare ad essere un investimento e cessare di essere un diplomificio. Il suo finanziamento perciò non può che essere commisurato al numero degli iscritti, ma anche complementare al contributo diretto delle famiglie, perché anche gli studenti vanno responsabilizzati ai loro doveri: studiare all'università è un privilegio-dovere di ogni studente, che costa non solo alla sua famiglia, ma a tutta la comunità che paga le imposte, anche a chi non ha figli. Se i contributi all'università fossero considerati un investimento e non una spesa improduttiva non dovrebbero essere tagliati così come è avvenuto. Il taglio ha infatti compromesso la competizione, l'organizzazione degli studi e soprattutto lo sviluppo della ricerca. Il ritratto impietoso fatto dalla Corte dei conti circa il fallimento del 3+2 ci chiama oggi tutti alla responsabilità di una riforma il più possibile condivisa e non più procrastinabile. Possiamo affermare che il disegno di legge n. 1905 pone i nodi strategici dello sviluppo del sistema universitario: in primo piano la *governance*, la struttura degli atenei, il premio al merito, la valutazione, lo stato giuridico dei docenti ricercatori e il loro reclutamento. L'obiettivo sembra essere quello di ridefinire in modo chiaro le regole del sistema, per creare un contesto che favorisca il pieno raggiungimento dell'autonomia. L'università deve infatti essere in grado di autoregolarsi al proprio interno, definendo un quadro generale di obiettivi strategici nazionali ed internazionali, con modalità di valutazione moderne ed efficaci, con la certezza dei premi, ma anche con la previsione delle sanzioni. Se parliamo di responsabilità, bisogna anche sanzionare la mancanza di responsabilità, quando questa è accertata. A nostro avviso la logica d'impresa può essere studiata e certamente presa in parte in prestito per la *governance* degli atenei, ma non trapiantata *tout poiché occorre invece introdurre procedure di governo del sistema più trasparenti, più veloci, più snelle e più finalizzate alla formazione culturale del capitale umano (che non è una materia inerte e pertanto non può essere assoggettata alle stesse regole che vigono nell'industria) e al progresso della ricerca, sia di base che applicata.

Riteniamo positivo l'aver valorizzato il ruolo del consiglio di amministrazione, in cui però i membri esterni devono essere nominati con precisi criteri che guardino soprattutto la competenza e l'esperienza e prescindano da qualsiasi intromissione della politica. Analogamente, il senato accademico deve certamente recuperare un ruolo più incisivo e più permeante le stesse scelte tecniche e amministrative del consiglio di amministrazione. Altrettanto positive riteniamo le novità che concernono il rettore e le sue competenze, come pure la novità degli accordi di programma, che consentono la sperimentazione di nuovi percorsi di tipo organizzativo, nonché quelle circa il reclutamento e lo stato giuridico dei docenti, in cui si registra la parziale eliminazione di alcuni automatismi e l'introduzione di valutazioni di merito e nuove regole concorsuali. Largamente condivisibile poi è l'esercizio dell'autonomia degli atenei nella scelta dei docenti sulla base di precisi criteri e di una idoneità nazionale, anche con il contributo di studiosi stranieri. In effetti, c'è il tentativo di uscire dal provincialismo in cui sono vissute per troppo tempo le nostre università, per aprirsi a livello internazionale e concorrere ad armi pari sul mercato del lavoro mondiale. L'autonomia deve essere applicata Se però l'autonomia significa anche responsabilità, non si può ritenere che sia indispensabile l'eliminazione del controllo da parte della Corte dei conti, perché la cosa confligge. Le norme che riguardano lo stato giuridico, che hanno visto eliminato l'obbligo delle 1500 ore, sono state modificate in modo più liberare e meno burocratico soprattutto per il regime delle incompatibilità. Rivolgiamo un plauso anche al relatore, che tanto si è prodigato per tutto il corso dei lavori. È ancora aperto, però, il problema dei ricercatori come quello delle università virtuose, che non possono non prevedere delle deroghe rispetto alle altre università proprio per l'impianto di tipo meritocratico della riforma stessa. Da sottolineare infine rispetto al personale è il blocco degli scatti stipendiali dei docenti, che è assolutamente inconcepibile, ingiustificato ed illegittimo e costituisce un elemento negativo volto a scoraggiare i giovani nei confronti della carriera universitaria. Poiché infatti gli scatti sono collegati al merito e non sono concessi più su una base di automatismo, sia i professori che i ricercatori debbono riottenerli al più presto (sarei contenta se avvenisse proprio nella fase in cui si discute la riforma), così come è avvenuto per i magistrati e per gli insegnanti. Il nostro Gruppo ha presentato numerosi emendamenti che spingono e sostengono scelte più incisive ed efficaci, come ad esempio quella dell'abolizione del valore legale del titolo di studio (a nostro avviso, riforma imprescindibile per un sistema formativo che è fondato sul merito, l'efficienza e l'efficacia) e molti altri emendamenti più tecnici e semplificativi dell'organizzazione ed altri sullo stato giuridico dei docenti. Valuteremo Valuteremo con responsabilità se il relatore ed il Governo sapranno apprezzarli. Il neo più forte di questo provvedimento resta comunque il suo inadeguato, o meglio inesistente, finanziamento.

pertanto, riteniamo che per il Governo sia un dovere costituzionale dare piena copertura alle nuove norme al fine di "dare gambe" ad una riforma che altrimenti resterà ancora una volta - noi non lo vorremmo - una riforma semplicemente sulla carta.

intervengo dopo che vari validi colleghi del Partito Democratico sono già intervenuti sull'argomento, e farò il tentativo di non ripetere le numerose osservazioni che ho condiviso. Per dare la dimostrazione del fatto che non parlerò a vantaggio di una visione del centrosinistra precostituita, sottolineo che il centrosinistra storico non ha motivi per vantarsi della propria azione sulla realtà universitaria: tutto perché anche il centrosinistra ha fatto mancare risorse significative nel passato (i tentativi del Governo Prodi sono stati lodevoli, ma in realtà insufficienti), e poi perché non ha fronteggiato molti motivi di difficoltà che ha avuto di fronte. Così, la moltiplicazione delle sedi di corsi di laurea ha disperso le risorse universitarie; l'ampliamento crescente delle fasce docenti superiori, e quindi il restringimento relativo della fascia dei ricercatori, hanno trasformato la forma della piramide universitaria

Hanno contribuito a rendere farraginoso il meccanismo anche l'attribuzione, peraltro inevitabile, di compiti didattici ai ricercatori, per coprire insegnamenti che non avevano copertura, la trasformazione fisiologica del ruolo dei ricercatori anche con i dottorati di ricerca, che ad un certo punto, per il fabbisogno dell'insegnamento, vanno ad intasarsi nell'imbuto della necessità della didattica.

Nella mia università, a Firenze, più della metà dei corsi è attivata con contratti a titolo gratuito. Detto tra noi, questa è una contraddizione in termini: che cosa potrà mai contrattare un ricercatore, una volta che ha sottoscritto un contratto a titolo gratuito?

dei corsi «3+2» costituiscono una preparazione semplificata, generica, in ciò stesso sta la difficoltà del passaggio ai due anni successivi di corso specialistico, perché chi arriva all'approdo, al corso specialistico, lo fa non sulla base di un cammino mirato a quell'obiettivo, ma sulla base di un cammino mirato a conseguire un diploma generico e spesso insoddisfacente.

Se ci troveremo nella condizione, tra breve, di importare insegnanti di matematica indiani, ciò dipende anche dal fatto che molti studenti italiani preferiscono la laurea in scienza delle comunicazioni e in psicologia e rifuggono dalla frequentazione delle scienze "dure". Di fronte a questo quadro molto problematico, di cui le responsabilità sono molteplici e non attribuibili a nessuna parte politica in particolare, il Governo ha esercitato un'azione nell'ambito del discorso pubblico e un'azione nell'ambito del discorso parlamentare. Come molti altri colleghi, riconosco ad alcuni membri della Commissione istruzione, in particolare al relatore, un'attenzione alla natura interna dei problemi; però, dal punto di vista

letteralmente micidiale delle risorse, tanto che le strutture universitarie sono sostanzialmente deprivate del minimo necessario per continuare ad andare avanti,

terreno comune, non di intesa, ma di confronto). In realtà, la scena pubblica del Popolo della libertà è stata saturata dall'idea di una lotta contro il baronato: insomma, il PdL si è presentato come forza progressiva che smonta il baronato. che smonta il baronato. Ora, dentro questa retorica pubblica c'è una strana aporia: è come se i baroni fossero tutti di centrosinistra

negli ultimi mesi abbiamo visto molti magistrati di centrodestra compromessi fino al collo in rapporti indicibili di tipo affaristico, rapporti curiosi o quanto meno degni di osservazione critica. Bisogna quindi vedere la prova dei fatti.

praticamente le fonti di alimentazione dell'università. In questo provvedimento, se non sarà cambiato con gli emendamenti, si dice ben 16 volte che gli interventi da realizzare sono senza oneri per lo Stato.

con la visione pluralistica che i colleghi della Lega vorrebbero esercitare attraverso la loro attenzione al federalismo. Esiste una tendenza centralistica nei confronti dell'autonomia universitaria, e dobbiamo vedere alla fine cosa ne verrà fuori. Sento di poter dire che, anche se esponenti autorevoli del centrodestra ogni tanto spezzano lance a favore dell'autonomia universitaria, in realtà quello che domina poi è un criterio di imperio centralistico. La questione del rapporto tra senato accademico e consiglio d'amministrazione forse è stata ridimensionata rispetto all'inizio quando c'era un totale predominio del consiglio d'amministrazione nei confronti del senato accademico che, in realtà, fotografa una filosofia aziendalistica: l'idea che c'è chi

Dentro questo corpo di cose molto problematiche, su cui si sono fatte scelte pesanti, c'è fondamentalmente l'inadeguatezza del reclutamento. A me sembra che si possa parlare, così come siamo ridotti oggi, di una sorta di università troncata. È la fine di un mondo. Forse per il centrodestra è positivo; a me fa venire in mente - se mi passate il paragone, che è il solo di tipo letterario che farò - la Sinfonia degli addii di Haydn, dove man mano che la sinfonia finisce gli orchestrali spengono la loro candela, si alzano e se ne vanno. Alla fine non resta più nessuno. Temo che nell'università pensata in questa maniera il troncamento decisamente brutale del corpo docente, con il blocco sostanziale del reclutamento,

e non solo, perché il mondo del lavoro è ormai totalmente dominato dall'insorgenza del precariato e, qualche volta, anche del lavoro non pagato.

Sembra che non tengano conto di un futuro possibile: verrà un giorno in cui tutte queste forze del precariato troveranno una forza per manifestarsi, un'intenzione! Ma non ci pensa nessuno. Oggi tutti considerano il precariato una forma plastica e mobile di gestione del lavoro, per cui chiunque deve essere prono alle esigenze del mercato, prestare la propria opera a basso prezzo e con scarse garanzie ed essere pronto a farsi fare fuori appena l'autorità superiore decide che così deve essere: entri ed esci dal mercato del lavoro in una forma che dipende dall'occasionalità, dalle ragioni di bilancio, dalla volontà di un consiglio d'amministrazione. Questo si vede tra l'altro, in parte, anche nei dipendenti irregolari del Parlamento, però, in confronto, questi sono dei privilegiati. Ci sono tutti gli altri che sono un esercito industriale di riserva, che con acume e serietà andrebbe visto in maniera diversa. Credo che nei confronti dei ricercatori, dei precari e dei dottori di ricerca un maggiore interesse verso la loro natura la loro natura di risorsa umana preparata sia d'uopo. Trovo che considerare "a perdere" una generazione di ricercatori confermati e determinare una situazione di incertezza per tutti i nuovi ricercatori significhi avere un atteggiamento indifferente alla ragione e al sentimento di chi si appresta a diventare soggetto di didattica e di ricerca. Chi si misura con questo lavoro non ha un grandissimo interesse per i soldi. Penso che la severità della selezione di mercato sia una cosa anche giusta nei confronti di chi compete duramente in un mercato vero, in cui la posta è diventare ricco, ricchissimo oppure no. Ma un soggetto, uomo o donna, che ha questa sorta di furiosa vocazione altruistica alla trasmissione della conoscenza ed alla stimolazione della curiosità per la ricerca non può essere trattato alla stessa stregua di un aspirante di un laboratorio di *broker* finanziari o di un tecnico della grande industria. Qui c'è una specie di forzatura: si immagina una forma di competizione, ma questo non è un libero mercato. Tutti voi sapete che il libero mercato in Italia è una finzione e che la concorrenza non esiste, e che, in particolare nel mondo

borse di studio ai meritevoli e bisognosi sono incerte; i prestiti d'onore scivolano pericolosamente verso la figura dell'indebitamento alla cieca. Come si fa a realizzare qualità senza investimenti? Qui ci viene detto che sostanzialmente la valutazione della qualità è fondamentale. Ma la qualità senza investimenti? L'ANVUR che c'è e non c'è?

è poi il problema interno della valutazione. La valutazione dei lavori scientifici e delle scienze "dure" è filtrata attraverso «*Science & Nature*», e il meccanismo dei *referees*.

allora per forza sei un genio. Spesso, nelle scienze umanistiche esistono meccanismi parcellari di discipline separate, collegate ma che fanno riferimento a mondi editoriali diversi. Non è facile. Qui mi sarebbe piaciuto che ci fossimo che ci fossimo posti il problema in maniera più approfondita. Penso che insomma - se devo dare una valutazione - anche adottando la logica del centrodestra che non condivido, questo provvedimento avrebbe potuto provare a costruire un po' di più, e soprattutto avrebbe dovuto rispondere ad un atteggiamento più problematico. Tra alcuni colleghi in Commissione io l'ho trovato; però alla fine il disegno di insieme non appare problematico, non appare interrogativo. Voi direte che si tratta di un provvedimento di legge che come tale però qui siamo di fronte alla necessità di una modificazione profonda. Forse sarebbe stato più giusto per il futuro, dovendo produrre uno sforzo di lungo periodo, che anche all'interno del centrodestra si incorporassero molti dubbi.

andranno verso un'onesta pensione e che i dipartimenti verranno fuori come protagonisti fondamentali. In conclusione, temo che si sia agli albori di una sorta di processo malthusiano di riduzione e

che in realtà non è veramente garantita, e in secondo luogo, la trasmissione della conoscenza, con tutto ciò che di problematico e critico ha dentro di sé, e dunque non una scienza di partito - per Giove! - ma la capacità di capire che il reale è complesso. la stimolazione e la curiosità della ricerca: se i ricercatori sono costretti a lavorare per niente e ad avvilirsi nell'inedia, è difficile riuscire a sviluppare nella società italiana la curiosità per la ricerca. Penso che di tutti i compiti fondamentali quello dell'istruzione alta sia proprio questo:

si possa superare questo momento, ma non trovo motivi di fiducia per vedere realizzato positivamente di questo disegno. Penso che di fronte a noi abbiamo un compito molto più vasto, al quale ci accingeremo.

saluto il Presidente) e in particolare al relatore, senatore Valditara, che ha svolto un lavoro certamente apprezzabile e prezioso. Vorrei sottolineare che questa circostanza non è frequente nella nostra Assemblea, e ricordo solo due

dalla maggioranza e che invece, come ben si vede, è stata immediatamente definita non inviolabile dai membri del Governo non appena approdata nell'altro ramo del Parlamento,

la qualità e, se posso dire così, la dignità del nostro lavoro parlamentare. Non tocca a chi, come me, siede nei banchi dell'opposizione qualificare la bontà del processo legislativo e dei suoi esiti (è un'opinione politica, ognuno di voi avrà la sua), la sua), ma come senatori della Repubblica possiamo mettere in rilievo il contributo del Senato della Repubblica. In questo caso penso si possa dire che la pagina che si è aperta con la discussione generale, e tra poco con tra poco con l'esame degli emendamenti, sia importante proprio per la vita del Senato, perché il Senato può trasformare quella che certamente era una riforma significativa in un testo di valore. Dunque, in questo caso il Parlamento e l'Assemblea fanno il loro dovere di organo legislativo, di ascolto delle posizioni e di costruzione delle soluzioni. Ora, è il caso di dare un giudizio sulla riforma senza darlo sulle risorse disponibili? Questo è un punto rilevante del dibattito che attraversa in particolare le forze dell'opposizione. Oppure dobbiamo dare un giudizio sulla riforma prescindendo dall'entità delle risorse disponibili? È evidente, signora Ministro, che le due cose si tengono, ma penso sia innanzi tutto utile giudicare

assolutamente indispensabile al nostro sistema universitario, e contiene elementi qualificanti di valorizzazione del merito e una capacità potenziale di far emergere i talenti, spesso inespressi nell'ambito del nostro sistema universitario. Nel corso della sua visita per l'inaugurazione della nuova sede della Scuola internazionale superiore di studi avanzati a Trieste, appena dieci giorni fa, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha fatto delle dichiarazioni molto impegnative che ci riguardano da vicino. Voglio essere chiaro: non amo l'uso strumentale delle parole del Presidente della Repubblica; il senso della sua funzione è quello di esercitare un compito che sia il meno possibile sfruttabile a fini di parte. Credo tuttavia si debbano interpretare, questa volta coerentemente, le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica a Trieste dell'utilità del nostro dibattito. Il Presidente ha detto ai ragazzi e ai docenti di Trieste: «Nessuno, anche e in modo particolare i giovani, di quanti operano e studiano nelle nostre università a qualsiasi livello può negare l'esigenza di una riforma. Noi abbiamo avuto, non nascondiamocelo, scelte discutibili e onerose, ad esempio di proliferazione delle sedi e di proliferazione dei corsi di laurea. Abbiamo avuto fenomeni di disordine e di inefficienza nella *governance* del nostro sistema universitario. A ciò deve porre riparo una legge di riforma che spinga il sistema universitario italiano verso livelli di produttività e di competitività sempre più alti nel rapporto con gli altri Paesi, europei e non soltanto europei». Ha detto poi il Presidente, e questo

lo voglio dire apertamente - che legge di riforma e dotazione adeguata di risorse per il funzionamento dell'università e della ricerca siano due facce della stessa medaglia».

tuttavia, le parole del Capo dello Stato non possono non interpretarsi nel senso che nel votare la riforma, nel dare il nostro giudizio sulla riforma, compito precipuo dell'Assemblea del Senato, non possiamo prescindere da quelle che ci attendiamo essere le dichiarazioni del Governo sulla possibilità di implementarla, di farla vivere attraverso

escludere una riorganizzazione del sistema universitario se contestualmente non sono appostate le risorse. Ma in ogni caso sarebbe impossibile prefigurare l'attuazione della riforma

dell'opposizione - dipenderà, in modo trasparente e laico, dall'esito dei voti dell'Aula e, dunque, dall'accoglimento di modifiche indispensabili.

le risorse necessarie per il comparto, per un importo stimato pari ad 1,3 miliardi di euro per il 2011, al fine di consentire il regolare avvio dell'anno accademico, di superare l'attuale grave crisi finanziaria del settore e di assicurare l'efficacia implementazione della riforma». Abbiamo presentato un numero limitato di emendamenti,

penso a quello che favorisce la mobilità interregionale di professori e ricercatori, penso a quello che consente agli assegnisti l'estensione della normativa sulla maternità e il congedo per malattia, penso a quello che incrementa le erogazioni liberali a favore di università ed istituti di istruzione universitaria, portandolo sino al 5 per cento. È infatti evidente che se vogliamo stabilire un rapporto virtuoso tra l'offerta e la e la domanda dobbiamo creare un meccanismo in base al quale il sistema dell'impresa possa investire sul mondo universitario in quanto esso fornisce la materia prima (laureati e specializzati) per la la domanda che il sistema produttivo esprime. Naturalmente gli emendamenti cruciali sono quelli che riguardano le risorse: ce ne occuperemo

Presidente, come si fa a riconoscere - come è avvenuto in occasione dell'ultima manovra economica - le prerogative degli insegnanti (come era doveroso), dei poliziotti di tante altre categorie quanto agli scatti di stipendio, e negarle proprio al mondo dell'università che si vuole legare ad una riforma così significativa? Lo stesso vale, naturalmente, per i ricercatori. Noi riteniamo che si debbano aprire delle finestre credibili

di chiamata. Ho usato l'espressione *senior track* e mi permetto di dire che invece c'è un nostro emendamento che propone di togliere la parola "*performance*"

penso che sia dovere e compito proprio del Parlamento lavorare per il miglioramento di un provvedimento così importante; penso sia compito e dovere politico di forze riformiste, di cercare di contribuire. La ministro Gelmini sa che, al termine di questo esame, potrà avere il voto di una componente dell'opposizione (una componente piccola, certamente, e che è e resta con chiarezza all'opposizione) se, e solo se, le riflessioni svolte dal Capo dello Stato fondamentalmente saranno accolte, ovverosia se sarà accolta la forte esigenza di legare questa riforma, su cui noi esprimiamo un giudizio

ha deciso di attuare tagli drastici, operando una riorganizzazione dei *Länder* tedeschi e un ridimensionamento della spesa per una serie di enti ritenuti non indispensabili in quel grande Paese, per destinare 20 miliardi di euro ai settori della ricerca e dell'università. Non ci aspettiamo questo, però sappiamo che una una riforma che certamente entra qui con limiti e difetti, che non è rivoluzionaria, che può essere una buona riforma ed è senz'altro migliorativa

signora Ministro, onorevoli colleghe e colleghi, il disegno di legge che giunge oggi all'esame dell'Assemblea si configura come un momento di singolare rilievo politico, in cui questo ramo del Parlamento è chiamato a svolgere un'opera di riordino e quindi un'azione riformatrice in materia di organizzazione delle università. Esso è il primo provvedimento corposo, organico, che riforma l'intero sistema dei nostri atenei e che punta ad affrontare in maniera seria e coraggiosa i problemi che esistono all'interno dell'università, nell'ottica di ridare maggiore peso ed autorevolezza

anche in seguito alle numerose audizioni, sottolineando il rilievo dei molteplici ed autorevoli interventi di senatori anche esterni alla 7a Commissione un dibattito di elevato tenore culturale, serio, pacato e approfondito, come peraltro dovrebbe sempre avvenire in Parlamento. In questo senso, mi preme anche evidenziare l'ampia coincidenza registrata fra maggioranza ed opposizione nella comune valutazione di molti punti decisivi del disegno di legge governativo, anche se su altri punti le difformità e le divergenze in parte rimangono. Nel registrare perciò positivamente il clima costruttivo che ha caratterizzato l'attività della Commissione, esprimo il mio più vivo compiacimento per la direzione intrapresa in favore della qualità della formazione universitaria, del rafforzamento dell'autonomia in un contesto di responsabilità, nonché della valutazione. Prima di entrare nel merito dei grandi temi che caratterizzano la riforma mi siano concesse una breve riflessione ed un'analisi di carattere generale relative alle sorti riservate alle tante riforme universitarie approdate in Parlamento. Il nostro Parlamento i cittadini italiani hanno una lunga e duratura consuetudine con le riforme dell'università: molte, per la verità, disperse ed abbandonate lungo i percorsi di più legislature; altre compiute, ma tutte unanimemente accolte - a torto o a ragione - con la critica che quel che si proponevano di realizzare era sempre o troppo o troppo poco. Troppo per chi è dell'avviso e resta convinto che le norme in un ambito così peculiare e specifico come quello degli atenei debbano solo tracciare il terreno su cui costruire l'edificio della autoregolamentazione delle università, lasciando all'autorità pubblica solo il compito di stabilire obiettivi di sistema, compatibilità economiche e strumenti di valutazione. Troppo poco per gli eterni scontenti, i quali ritengono che, naturalmente, «ci vorrebbe ben altro» per imporre un vero salto di qualità, cioè finanziamenti a pioggia agli atenei, indipendentemente dalle loro capacità di sviluppo e di produzione scientifica e culturale. Sarebbe, quindi, un vero peccato se tale rituale si ripetesse anche per questo nuovo provvedimento di riforma dell'università italiana, una volta licenziato dal Parlamento per essere destinato a diventare operativo nella sua concretezza. Sarebbe un peccato perché questo provvedimento governativo, fortemente voluto dalla ministro Gelmini e approdato al vaglio dell'Assemblea dalla 7a Commissione del Senato, propone nel suo complesso un decisivo passo avanti in un settore la cui crisi d'identità, anche anche se talora esagerata e strumentalizzata all'esterno da alcune frange irresponsabili dell'opposizione politica, è comunque sotto gli occhi di tutti. Le analisi delle origini della crisi delle nostre università non possono certamente accontentarsi di scavare nel nostro più recente passato. Pensare, difatti, che la crisi nasca con la riforma del «3 più 2» o che si possa racchiudere in essa significherebbe accontentarsi di una lettura distratta di almeno 40 anni di provvedimenti, spesso nati sull'onda dell'emergenza, spesso causa a loro volta di emergenze future, quasi mai collegati tra loro da una visione d'insieme. Obiettivo di quella riforma, approvata nel 2000 da un Governo di centrosinistra, era quello di rendere più standardizzati, brevi e flessibili i percorsi didattici dei vari corsi, con finalità direttamente collegate all'esigenza di avere un maggior numero di iscritti all'università: dunque, più laureati e con maggiori possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro rispetto a quelle prospettate dall'istruzione superiore in passato. I risultati? Sono sotto gli occhi di tutti: un fallimento. Le sedi? Troppe, come i professori. Gli studenti? Molti i fuori corso e pochi i preparati. I costi? Insostenibili. Le università? Troppe. onestà intellettuale vuole di dichiarare anche che non sta lì l'origine della crisi, ma in vari decenni di provvedimenti di emergenza. con urgenza, di mettere in chiaro alcune regole fondamentali. La prima, per esempio, è che l'autonomia delle università, di cui a volte si parla a sproposito, intanto è un valore in quanto è usata bene; e, se non funziona, è necessario accompagnarla con criteri di qualità accademica e regole finanziarie che impediscano ulteriori degenerazioni. La seconda è che le università devono elaborare programmi e progetti ed essere valutate e finanziate a seconda di come li realizzano, anziché navigare a vista cercando di fare tutte di tutto e di più. Non ha senso imporre centralmente, a priori, missioni diverse per le diverse istituzioni, ma è indispensabile chiedere a ciascuna di concentrare le energie su quanto pensa di poter fare meglio e con maggior profitto per la collettività. Quasi 300 sedi, migliaia di corsi di laurea, oltre 2.000 corsi di dottorato: sono numeri che fotografano una deriva dell'apparato universitario italiano, non una vera espansione organica del sistema. Esigere dunque che l'ampliamento dell'offerta - in qualche misura naturale e giusto prodotto della trasformazione, incompiuta e imperfetta, di un sistema per pochi in un sistema per molti - sia ripensato nel rispetto di standard qualitativi elevati elevati è uno degli obiettivi prioritari che il provvedimento odierno si propone di raggiungere. L'autonomia, pertanto, la valutazione, la responsabilizzazione degli atenei dal punto di vista gestionale, scientifico e didattico; una *governance* snella ed efficace; un criterio di reclutamento in linea con la migliore prassi internazionale diventano in questo senso l'asse dell'intero sistema. Sarebbe però illusorio pensare che nuove modalità di valutazione della ricerca e della didattica, per quanto incisive, producano dall'oggi al domani effetti taumaturgici. L'esperienza dei Paesi da tempo impegnati in questa direzione, come la Gran Bretagna, insegna che ci vuole almeno qualche anno perché la valutazione riesca a permeare i comportamenti e le scelte dei singoli e delle istituzioni. in un sistema compiutamente orientato sull'asse autonomia-valutazione non servirebbe richiedere l'abilitazione scientifica per chi aspira a un posto da professore. Prevedere, perciò, almeno per qualche anno, che le università siano libere di scegliere i propri docenti tra quanti hanno superato questa preselezione a livello nazionale costituisce oggi il punto di mediazione più spinto tra chi aspira a un sistema del tutto liberalizzato e chi ne teme la dequalificazione definitiva. Non è un caso che su questo elemento decisivo si sia registrata in più punti piena convergenza tra maggioranza e opposizione. In tale ottica, ritengo, il testo predisposto dalla Commissione, pur essendo perfettibile, ha comunque raggiunto un buon risultato, senz'altro migliorato dall'approvazione di emendamenti di estrema ragionevolezza presentati da entrambi gli schieramenti. Il destino di una legge di riforma universitaria, com'è noto, dipende molto dalle risposte che sarà in grado di dare, soprattutto a quanti aspirano a dedicarsi alla ricerca universitaria, ai ricercatori e agli associati in servizio, che non solo non hanno beneficiato della riforma del 1998, ma cui anzi essa ha sbarrato la strada. Qui, allora, l'alternativa è secca: o riproporre una soluzione demagogica come quella già esperita, con risultati catastrofici, almeno tre volte negli ultimi quarant'anni, facendo esplodere gli organici con *ope legis* e immissioni in massa di ruolo, o disegnare un sistema rigoroso che finalmente distingua tra reclutamento e progressione di carriera interna senza annacquare i requisiti scientifici, ma garantendo a ciascun docente il fondamentale diritto ad essere valutato con tempi certi e modalità serie. Il fatto che la gran parte dei ricercatori, degli associati e dei precari invochi oggi criteri qualitativi rigorosi, non scorciatoie, lascia sperare che forse qualcosa potrà davvero cambiare per il meglio. In particolare, a questo proposito, vorrei ricordare che sono state introdotte norme a tutela dei ricercatori a tempo indeterminato, trascurati dal testo originario, e che passi ulteriori potranno essere compiuti in Aula. Con l'attività emendativa, per esempio, è stato riequilibrato il rapporto tra senato accademico e consiglio di amministrazione, di cui è stato peraltro fissato il numero minimo di componenti esterni, che in molti casi finiranno - spero di no! - per essere addirittura inferiori rispetto al contesto attuale. Assieme a questi temi non vorrei tralasciare una brevissima riflessione sugli attuali modelli maggiormente in uso nei sistemi universitari stranieri. In Francia, Germania, Italia e Spagna vige il modello europeo tradizionale, con un'autonomia piuttosto limitata e in cui il controllo interno è prevalentemente affidato ai docenti. Negli Stati Uniti d'America gli atenei pubblici e privati sono fortemente autonomi, ma il controllo è essenzialmente esterno. Nei Paesi anglosassoni, invece, gli atenei sono fortemente autonomi e negli ultimi decenni il controllo si è spostato da un sistema di sostanziale autogoverno dei docenti a un modello molto vicino a quello americano. In altri Paesi, tra cui Svezia, Olanda, Austria, Danimarca e Giappone, si è passati dal modello tradizionale europeo a una forte autonomia con una *governance* di tipo americano. Il modello italiano, ovviamente, si configura come un modello *sui generis* dove, in particolare, il potere decisionale è in capo ai docenti dell'ateneo, con conseguente forte autoreferenzialità. Molte decisioni sono pertanto prese sotto la spinta di interessi interni corporativi, mentre gli obiettivi istituzionali più generali passano in secondo piano. Le cariche sono prevalentemente elettive, mentre il potere decisionale finale è quasi sempre assegnato ad organi collegiali, sicché la responsabilità formale individuale è piuttosto limitata. Si tratta, in sostanza, di poteri "politici", basati essenzialmente e soprattutto sulla capacità di acquisire consenso. Recentemente ho avuto modo di approfondire la riforma universitaria austriaca del 2002, che ha potenziato l'autonomia degli atenei e ne ha completamente modificato la *governance*, realizzando un modello intermedio più vicino a quello anglosassone. il disegno di legge del Governo riprende in buona sostanza, in modo complessivamente coerente, buona parte delle misure già introdotte con successo nei sistemi universitari dei principali Paesi dell'OCSE. Un altro degli obiettivi essenziali cui esso tende è quello di riformare l'università fuoriuscendo dalla cultura dell'emergenza, la quale può avere solo una natura contingente e una durata limitata, mentre in una riforma organica bisogna delineare il futuro dell'università italiana, onde evitare che il prossimo e futuro Governo ricominci tutto daccapo. Il provvedimento del Governo ha il merito di proporre un modello organizzativo che contempera il rispetto dell'autonomia universitaria con le responsabilità che ne derivano. L'approccio organico del progetto di legge governativo procede insomma ad una riforma complessiva e a tutto campo dell'università, di cui sicuramente si sentiva l'esigenza. Nel dibattito in Commissione è emersa l'esigenza di raccordare meglio didattica e ricerca, attraverso una rinnovata centralità dei dipartimenti, di semplificare le strutture decisionali e di favorire la collaborazione fra società e università, anche in un'ottica di riequilibrio delle opportunità connesse al diverso tessuto territoriale nazionale. In questo senso, il provvedimento costituirà - ritengo - una valida soluzione per porre fine a varie patologie che, soprattutto in quest'ultimo periodo, hanno afflitto le università, quali ad esempio le deleterie e dannose deviazioni corporative, un reclutamento del corpo docente non sufficientemente attento alla qualità, l'eccessiva moltiplicazione delle sedi e, spesso, sprechi di finanza pubblica. una grande riforma, molto impegnativa, che trova il suo equilibrio tra modello continentale e quello americano, con prevalenza del modello europeo. In questo quadro organico di riordino, e quindi di un'azione riformatrice in materia di organizzazione delle università, è possibile ritenere che, in una prospettiva di breve periodo, potranno essere ridotte le sedi esistenti, anche facendo leva sullo strumento della fusione o della federazione, al fine di concentrare i fondi, garantendo selezione e competizione al rialzo verso le eccellenze.

di un codice etico, per evitare incompatibilità e conflitti di interessi legati a parentele; alle università che assumeranno o gestiranno le risorse in maniera non trasparente saranno ridotti i finanziamenti

Il senato avrà compiti di indirizzo e avanzerà proposte di carattere scientifico, ma sarà il consiglio di amministrazione ad avere la responsabilità chiara delle spese, delle assunzioni e delle spese di gestione anche delle sedi distaccate. sarà fortemente responsabilizzato e competente. Ci saranno una presenza qualificata degli studenti negli organi di governo e un nucleo di valutazione d'ateneo a maggioranza esterna. Anche gli studenti avranno finalmente la possibilità di valutare i professori. Vi sarà, inoltre, la possibilità per gli atenei di fondersi tra loro o aggregarsi su base federativa, per evitare duplicazioni e costi inutili. riduzione dei settori scientifico-disciplinari, la riorganizzazione interna degli atenei, l'abilitazione nazionale e la chiamata diretta degli abilitati con assunzione di responsabilità di chi assume. di chi assume. Si pone infine il problema di ripensare le modalità di attribuzione delle risorse, che indubbiamente vanno correlate anche ai risultati, atteso che le disposizioni sul reclutamento e sulla *governance* configurano una riforma di sistema e, pertanto, non necessitano di finanziamenti. Ma indubbiamente il problema dei finanziamenti e delle risorse si pone, anche se sotto altri aspetti. Va ricordato intanto che nel 2010 il taglio di 672 milioni previsto si è ridotto di oltre la metà, grazie ai 400 milioni recuperati alla fine dello scorso Si tratta di una decurtazione senza dubbio dolorosa, ma sopportabile se confrontata anche con quanto è accaduto in altri Paesi. Si tratta allora di riorientare la spesa sul diritto allo studio e sulla qualità della ricerca, evitando gli sprechi verificatisi negli ultimi anni e non certamente ascrivibili alle riduzioni di risorse operate dal Governo. Non voglio qui menzionare la drammatica situazione in cui versano alcune università italiane, cui presumibilmente se ne aggiungeranno altre, ma va detto che si tratta di situazioni comunque dettate non dalla riduzione del FFO bensì da errori accumulati nel tempo e oggi non più sostenibili. Errori non tanto da deplorare, quanto piuttosto, in assoluto, da condannare. Come vanno, senza eccezione alcuna, condannate le assunzioni fuori controllo, le gestioni mirate ad acquisire il consenso e le promozioni senza copertura: errori, questi, che hanno registrato nell'ultimo decennio un incremento del corpo docente pari a circa il 24 per cento nonostante una sostanziale parità di studenti, per non parlare, oltre a ciò, di un aumento dei professori ordinari di circa il 46 Rimane fermo in ogni caso l'impegno del Governo, come ha assicurato la stessa ministro Gelmini, del recupero di una parte delle risorse decurtate, al quale si farà fronte attraverso un tavolo tecnico incaricato di individuare le misure necessarie per mantenere le borse di studio e sostenere le spese correnti. Nell'esprimere perciò l'apprezzamento per il provvedimento di riforma universitaria proposto dal ministro Gelmini auspico che sia rapidamente approvato dalle due Camere con tutti i miglioramenti possibili che renderanno l'università italiana improntata non solo alla meritocrazia e alla trasparenza, ma ne faranno un volano per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.

dai banchi dell'opposizione, a lasciare da parte per un attimo il problema delle risorse, perché è un po' il *Leitmotiv* di tutti gli interventi svolti dai rappresentanti dell'opposizione. Vorrei concentrarmi sui temi emersi e le altre criticità sollevate. Devo dire subito, e l'ho notato con piacere, che all'interno dell'opposizione sono affiorati accenti molto diversi; ad esempio, il senatore Rutelli ha sostanzialmente apprezzato la riforma che stiamo discutendo in questo momento in Aula e devo dire che anche la senatrice Sbarbati, al di là di alcune critiche, ha dato una rassegna ampiamente positiva di alcuni dei punti qualificanti di questa nostra riforma. Quali sono allora negativi maggiormente sottolineati dall'opposizione? Anzitutto, è emerso il problema del ruolo del consiglio di amministrazione rispetto a quello del senato accademico. Devo dire subito che, da questo punto di vista, oggettivamente siamo su posizioni differenti:

i pareri, le proposte, i suggerimenti del senato accademico: deve tenerne conto, non può prescinderne. Credo che questo sia senz'altro un elemento importante per qualificare positivamente il ruolo del senato accademico.

al tema dei ricercatori a contratto e della sorta dei ricercatori a tempo indeterminato. Colgo certamente con forte sensibilità le preoccupazioni però devo anche aggiungere che noi abbiamo dato alcune risposte sia nel testo approvato in Commissione, sia, in particolare, negli emendamenti che, come relatore, ho presentato per l'Aula. Voglio citare, per esempio, fra questi emendamenti, quello che prevede l'obbligo di coprire nei prossimi sei anni posti da associato pari ad almeno un quarto dei ricercatori in servizio. Questa è una risposta molto forte che, in qualche modo, era stata sollecitata anche dalle organizzazioni dei ricercatori.

quello che diciamo nel testo del nostro disegno di legge dia sostanzialmente una risposta senz'altro positiva a questa preoccupazione e, d'altro canto, gli uffici mi hanno confermato questa interpretazione. Prevedere, Prevedere, infatti, un "obbligo ad assicurare la disponibilità delle risorse necessarie all'interno della programmazione, in caso di esito positivo della procedura di valutazione dei ricercatori a contratto", al fine di poterli

noi adottata consente di fornire una maggiore flessibilità organizzativa alle università, ma il risultato è sostanzialmente identico. È emerso negli interventi, ma soprattutto negli emendamenti che sono stati presentati dall'opposizione, il tema della terza fascia. Sono sostanzialmente contrario, come anche il Ministro, sostanzialmente contrario, come anche il Ministro, a questa ipotesi perché, nel momento in cui si mette ad esaurimento la figura del ricercatore a tempo indeterminato e nel momento in cui si introduce

o questi ricercatori hanno i titoli per poter conseguire un'abilitazione aperta ad associato o non li hanno; in questo caso, bisognerebbe riconoscere che si crea una figura una figura di minor livello, del tutto impropria, senz'altro più debole scientificamente della figura di professore cui si chiede la maturità scientifica. Bisognerebbe immaginare che per questi professori di terza fascia non ci sia ancora una piena maturità scientifica. Va anche aggiunto che, sebbene la grande maggioranza dei ricercatori insegnano, non tutti sono stati considerati idonei all'insegnamento. Se dovessimo immaginare una trasformazione *d'emblée* di tutti i ricercatori in professori di terza fascia, dovremmo immaginare una moltiplicazione dei corsi di laurea e una sorta di promozione *ope legis* anche per quelli Con riferimento al reclutamento sono rimasto perplesso di fronte ad alcune obiezioni avanzate da esponenti dell'opposizione e, in particolare, del Partito Democratico che hanno firmato il testo proposto che è sostanzialmente affine, soprattutto per quanto riguarda l'abilitazione nazionale, al nostro disegno di legge. Ho trovato un po' curioso che si facessero facessero delle critiche anche ingenerose a questo nuovo sistema di reclutamento soprattutto da parte di quei senatori che hanno firmato un testo che prevede il modello francese perché di questo si tratta.

del valore legale un effetto taumaturgico. Nel privato già oggi non c'è il valore legale, perché un'impresa assume non certo per il fatto che c'è un pezzo di carta;

in prospettiva si potranno fare dei passi avanti. Un primo passo avanti lo delinea già questo disegno di legge con l'accreditamento, che è la premessa per poter poi arrivare eventualmente ad un'abolizione del valore legale.

Abbiamo detto più volte che il testo che ci è pervenuto dal Governo peccava di un eccesso di centralismo e rigidità. Credo che in Commissione abbiamo raggiunto un buon equilibrio. Mi rendo conto che l'*optimum* (ne parlavo stamattina

veniamo anche da un periodo storico in cui le università hanno indubbiamente abusato dell'autonomia: abbiamo citato il caso di Siena, ma potremmo citarne tanti altri. Abbiamo vissuto

raggiungono dei risultati decorosi, ma manca un sistema di eccellenza. Per quanto riguarda l'eccellenza degli studenti, vorrei essere chiaro anche rispetto ad alcune interpretazioni giornalistiche: non sono per nulla d'accordo

ai ragazzi che raggiungano risultati di eccellenza. Infatti, badate che le borse di studio servono per garantire il successo formativo di quei ragazzi che provengono dai ceti sociali più disagiati il nostro sistema universitario è fortemente penalizzante sotto il profilo della promozione sociale. Se dovessimo immaginare ‑ come qualcuno propone ‑ di eliminare la garanzia di borse di studio assegnate in

quello che si è fatto in Germania e che si sta facendo ora in Francia: premiare i dieci dipartimenti migliori e le dieci università migliori, proprio per concentrare risorse straordinarie sul tema dell'eccellenza. Vorrei poi soffermarmi ancora su qualche tema che credo sia importante.

Credo che la risposta giusta sia invece quella di trovare delle risorse adeguate e di eliminare alcuni meccanismi penalizzanti, perché il vero problema dei nostri ricercatori non è tanto nei meccanismi

voglio dire con grande chiarezza - perché un ricercatore oggi entra in ruolo mediamente all'età di 35 anni: 35 anni: è evidente che se noi dovessimo immaginare che questo ricercatore, diventato professore, vada in pensione a 65 anni, ridimensioneremmo di molto le sue aspettative pensionistiche rispetto agli altri lavoratori

esprime un poco la disinformazione che su questo disegno di legge si ritrova spesso sugli organi di stampa. Un autorevole editorialista, Tito Boeri, ha sottolineato come

ritornate le facoltà, mentre sarebbero stati soppiantati i dipartimenti: peccato però che, proprio in Commissione, abbiamo eliminato nelle procedure di assunzione dei futuri professori il ruolo delle facoltà.

relativamente al discorso delle risorse. È inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Nella manovra finanziaria di questo autunno dovranno essere ridate risorse importanti e significative all'università italiana per consentire a questa ottima riforma di funzionare fino in fondo

una nuova finestra"). La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche al Calendario corrente e il nuovo Calendario dell'Assemblea fino al 4 agosto. I lavori di questa settimana saranno dedicati alla discussione del disegno di legge di riforma universitaria, al fine di pervenire auspicabilmente al voto finale entro la seduta pomeridiana di giovedì 29 luglio, per la quale non è previsto 1'orario di chiusura. Le votazioni degli emendamenti inizieranno domani mattina, a partire dalle ore 9,30 non appena pervenuto il parere della Commissione bilancio. Per quanto riguarda il disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza stradale,

Il Parlamento in seduta comune è stato riconvocato domani alle ore 12,30. Voteranno per primi gli onorevoli deputati. La chiama dei senatori avrà inizio intorno alle ore 14. Ove non si raggiunga un risultato positivo, è stato convenuto di indire ulteriori convocazioni anche a distanza ravvicinata, al fine di consentire nel più breve tempo possibile l'elezione di otto componenti del Consiglio superiore della magistratura. I lavori dell'Assemblea riprenderanno lunedì 2 agosto dalle ore 17 alle ore 21. Sono inoltre previste sedute martedì 3 e, se necessario, mercoledì 4 agosto con inizio alle ore 9,30 e con eventuale prosieguo nel pomeriggio, previa sospensione tra le ore 14 e le ore 15. La prossima settimana, oltre all'eventuale seguito di disegni di legge non conclusi, saranno discussi il decreto-legge recante proroga di missioni internazionali, il disegno di legge concernente il piano straordinario contro le mafie, già approvato dalla Camera dei deputati, ratifiche di accordi internazionali e documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Nella giornata di lunedì prossimo tornerà a riunirsi la Conferenza dei Capigruppo per definire il calendario dei lavori dopo la sospensione per la pausa estiva. **Programma dei lavori Signora Presidente, onorevoli senatori, ho ascoltato con grande interesse il dibattito sulla riforma universitaria. Si è compiuta oggi, infatti, una tappa fondamentale del cammino avviato ormai quasi due anni fa con le linee-guida sull'università cui hanno fatto seguito analisi, dibattiti e approfondimenti commisurati all'importanza della materia e alla complessità del disegno di legge. Si tratta infatti di un disegno di riforma organico che per la prima volta affronta il problema del reclutamento nel contesto di una riforma più generale dei meccanismi di governo, gestione e organizzazione degli atenei. La sua forza è proprio l'organicità. Per la prima volta da molti decenni il Governo e il Parlamento hanno l'occasione di offrire al nostro sistema universitario un modello compiuto e coerente, disegnato non in base a pregiudizi ideologici o ad irrealistiche fughe in avanti, ma basato su analisi ampiamente condivise dei problemi dell'università e maturato dalla consapevolezza che è venuto il momento di dare risposte concrete ai problemi annosi penso al tema dell'autonomia, a come coniugarlo con la responsabilità, ad una programmazione adeguata, ad una politica vera di diritto allo studio, per citare solo alcuni temi. Lo ribadisco: cerchiamo di muovere il ragionamento su un tema così delicato, non da un'ottica squisitamente politica, ma sapendo che l'università è un bene di tutti e la sua organizzazione deve obbedire ad una logica il più possibile condivisa, anche per garantire una ragionevole continuità nel tempo delle disposizioni normative. Diamo allora seguito all'invito del presidente Napolitano, che ringrazio ancora una volta per la costante attenzione che dedica al mondo dell'università e della ricerca. è stato ricordato poc'anzi dal senatore Rutelli, nel discorso tenuto a Trieste il 13 luglio il Presidente ha adoperato parole importanti. Ha detto: «Ci sono alcuni problemi, ci sono alcune scelte

7a Commissione ha svolto un grandissimo lavoro e in tal senso voglio ringraziare il presidente Possa, il relatore, senatore Valditara, e tutti i componenti della Commissione, che hanno partecipato ai lavori con grande impegno e riservando a questo tema il peso che merita. Da parte mia ho valutato con attenzione gli emendamenti presentati e intendo esprimere un parere favorevole su tutti quelli che siano in grado di contribuire a rafforzare l'impianto riformista e meritocratico del provvedimento. Il nostro sistema universitario vive - non certo per la prima volta - una fase difficile. L'analisi dalla quale sono partite le linee guida e le proposte del Governo non lascia molto spazio all'ottimismo. Abbiamo di fronte un sistema che, in molti casi, sembra aver perso la bussola, aver scambiato l'autonomia per licenza; un sistema che troppo spesso ha pensato a sé stesso e non alle esigenze dell'Italia. Soprattutto, il prestigio e la considerazione del Paese verso il mondo universitario sembrano, almeno in parte, offuscati. Troppo spesso le università occupano le pagine dei giornali più per gli scandali che per le scoperte, mettendo a rischio la legittimazione stessa di istituzioni che dovrebbero piuttosto essere prese a modello. L'amarezza di queste riflessioni è accentuata, non temperata, dalla constatazione che nei nostri atenei, giorno dopo giorno, operano con impegno e con ottimi risultati molti professori e ricercatori di alto valore, sinceramente dedicati al progresso della scienza e al bene comune, e studenti che desiderano acquisire nuove competenze e strumenti per il loro futuro. È soprattutto a queste persone che abbiamo il dovere di garantire un futuro all'altezza delle loro aspettative. Ed è proprio pensando a loro che dobbiamo cogliere questa opportunità di intervenire con decisione sui problemi dell'università, senza cercare di nasconderne o sminuirne la portata, ma avanzando soluzioni innovative e, se serve, drastiche. Vorrei anche sviluppare il tema dell'autonomia nonché cercare di rispondere ad una critica che viene mossa spesso ad questo disegno di legge, cioè l'accusa di essere dirigista. È certamente un'accusa facile, ma a mio modo di vedere ingiusta, perché le nostre università - non possiamo dimenticarlo - sono enti pubblici gestiti sulla base delle leggi in materia. Tutto va normato per legge: strutture di governo, diritti e doveri dei professori, meccanismi concorsuali, diritto allo studio, norme contabili. In questo contesto abbiamo compiuto ogni sforzo per snellire, semplificare e delegificare, anche grazie al contributo della 7a Commissione, che voglio ancora ringraziare. Oltre non è possibile andare e, in effetti, mi sembra che anche alcune proposte dell'opposizione si muovano all'interno dello stesso perimetro concettuale. Certo, personalmente sogno un futuro in cui la forza della valutazione e il suo impatto pervasivo sui comportamenti dei singoli e delle istituzioni consentano di abbandonare molte delle regole che oggi riscriviamo. Me lo auguro, ma non credo di peccare di pessimismo se affermo che i tempi per questa rivoluzione oggi non sono ancora maturi. Nel frattempo, invito gli onorevoli senatori a considerare con particolare attenzione le norme che già si spingono in quella direzione: penso alla possibilità che gli atenei virtuosi sperimentino proprie modalità di organizzazione e di gestione; alla facoltà data agli atenei medi e piccoli di semplificare ulteriormente la struttura interna, una norma che riguarda oltre la metà di tutte le istituzioni universitarie; all'eliminazione di macchinose procedure elettive per la formazione delle commissioni di concorso e alla completa libertà data agli atenei di regolare come meglio credono le procedure interne di chiamata, di selezione e di promozione. Intendo ora sviluppare alcune considerazioni più dettagliate su due punti che forse sono i più delicati della riforma: mi riferisco alla posizione dei ricercatori e alle questioni legate al finanziamento del sistema. Sono consapevole della situazione di disagio in cui versano gli attuali ricercatori di ruolo, che non a torto lamentano un ritardo trentennale della politica nel definire chiaramente la loro funzione e i loro compiti. La figura del ricercatore nacque nel 1980 senza che venissero definiti con la necessaria chiarezza le sue funzioni e il suo stato giuridico. Gli interventi successivi non hanno fatto che complicare questo quadro, già di per sé incerto. Oggi, cinque anni dopo che il ruolo è stato dichiarato ad esaurimento, anche se a decorrere dal 2013, occorre prendere atto con realismo e onestà intellettuale che le soluzioni possibili sono due e soltanto due. Possiamo proporre una qualche forma di *ope legis*, esplicita o mascherata, generosa o a costo zero, ma insomma un meccanismo che prescinda dalle normali regole di avanzamento in carriera. Si tratterebbe della riedizione di vecchie pratiche discreditate che hanno provocato guasti duraturi nel nostro sistema universitario e per le quali non si sente davvero alcuna nostalgia: non è infatti con altri provvedimenti errati o antimeritocratici che si può rimediare agli errori commessi in passato. Prendo atto con sincera soddisfazione e ammirazione che a non spingere in questa direzione è stata prima di tutto proprio la gran parte dei ricercatori, i quali chiedono di essere valutati singolarmente per i propri meriti e di non venire accomunati in un provvedimento collettivo che di fatto ne svilirebbe il Senato non pare intenzionato a proporre soluzioni di questo tipo. La seconda opzione è la più difficile, ma anche, ne sono convinta, la più onesta dal punto di vista scientifico e politico. Il disegno di legge introduce per la prima volta nel nostro Paese una chiara distinzione tra reclutamento e promozione. Per diventare associati o ordinari si deve conseguire un'abilitazione scientifica nazionale che consente di partecipare a rapide procedure di selezione bandite da ciascuna sede. Questa è, a mio modo di vedere, la via maestra che, anche a regime, regolerà un momento fondamentale nella vita degli studiosi. Si tratta di un meccanismo molto simile a quello francese, vicino anche a quello in uso nei sistemi anglosassoni, dove l'abilitazione non viene assegnata da una Commissione nazionale ma coincide di fatto con l'esito positivo di una consultazione di esperti esterni all'ateneo che garantiscono appunto l'idoneità dei candidati a monte della decisione locale. Su questo schema di fondo, ampiamente condiviso, abbiamo innestato specifiche previsioni per consentire che nei prossimi anni si possa dare un risposta concreta alle aspettative dei molti ricercatori che attendono di vedere riconosciuti i propri meriti. Prevediamo quindi che nei primi sei anni gli atenei possano chiamare a un ruolo superiore gli studiosi già in ruolo nell'ateneo stesso, con procedure particolarmente rapide e snelle, fino alla metà dei posti disponibili, sempre però a valle dell'abilitazione nazionale. A tal fine intendiamo operare per assicurare che nei prossimi anni una quota specifica del Fondo di finanziamento ordinario che dovrà essere integrato

Ai ricercatori, in modo particolare a quelli più giovani, chiedo quindi di valutare con serenità e realismo la proposta contenuta nel disegno di legge, quella di un percorso concreto per rimettere in moto un sistema ingessato. Faccio appello al loro senso di responsabilità per evitare che la protesta, sempre legittima, non si traduca in un grave danno per gli studenti. Dobbiamo renderci conto tutti che non esistono soluzioni miracolistiche, ma solo sforzi tenaci e e inevitabilmente graduali per raddrizzare le storture che si sono sedimentate negli anni. Per quanto riguarda il tema dei fondi, so bene che questo meccanismo funziona se ci sono le risorse per bandire i concorsi e, in generale, se il Fondo di finanziamento ordinario si mantiene a livelli più o meno costanti. Pertanto, occorrerà un impegno di tutto il Governo, così come è stato ribadito in sede di approvazione della manovra Da quando ho assunto la responsabilità del mio Dicastero mi sono battuta senza sosta perché, pur in un quadro molto serio di riduzione della spesa pubblica, il settore universitario venisse toccato il meno possibile. È doveroso ricordare che il Fondo di finanziamento ordinario per il 2009 è stato superiore dell'1 per cento a quello del 2008, nonostante il deteriorarsi del quadro macroeconomico. Con la legge n. 1 del 2009 abbiamo recuperato per il periodo 2009-2012 oltre 300 milioni di euro per il *turnover*, 135 milioni per il diritto allo studio e 65 milioni per gli alloggi e le residenze universitarie. Sono riuscita a far fronte alla promessa fatta dal mio predecessore e a finanziare, per 40 milioni di euro nel 2008 e 80 nel 2009, nuovi posti da ricercatore, anche se, sia chiaro, ho dovuto trovare *ex novo* quei fondi. Per il 2010 il taglio previsto originariamente era di 672 milioni di euro; quel taglio si è ridotto a meno della metà grazie ai 400 milioni di euro recuperati in finanziaria. Il Fondo di finanziamento ordinario per il 2010 sconta quindi una riduzione di circa il 3,7 per cento: riduzione dolorosa, certo, ma oggettivamente sopportabile. Anche quest'anno, nonostante la riduzione, distribuiremo poco più del 7 per cento dei fondi sulla base di un modello valutativo. Come Ministro dell'università sono naturalmente la prima a volere e a chiedere con forza fondi e investimenti. Ho però anche il dovere e, consentitemelo, lo abbiamo tutti, di guardare in faccia la realtà. Le cifre del dissesto sono impressionanti. Ora che abbiamo imposto maggiore trasparenza e serietà nella redazione dei bilanci stanno emergendo sofferenze troppo a lungo sottaciute che rivelano anni di diffusa irresponsabilità, di spese facili, di assunzioni fuori controllo, di promozioni senza copertura, di gestioni mirate ad acquisire il consenso dimenticando responsabilità e qualità. Dal 1999 al 2009 gli studenti sono cresciuti del 7 per cento, ma il corpo docente è cresciuto del 24 passando da 50.700 unità di ruolo a 62.700. Solo il costo di questi 12.000 nuovi docenti pesa per oltre un miliardo su un Fondo di finanziamento ordinario di 7,5 miliardi. Nello Nello stesso decennio, poi, il numero dei professori ordinari è cresciuto del 46 per cento, con punte del 70-80 per cento di crescita in alcune aree disciplinari. Molte università hanno dato corso alle chiamate ad un ruolo superiore ignorando intenzionalmente i maggiori costi che si verificano dopo il triennio di conferma, costi certi e ineludibili. Nel complesso quindi il costo degli stipendi è lievitato da 4,5 a 6,8 miliardi, con un aumento di 2,3 miliardi, il 51 per cento in più rispetto a dieci anni fa. Oggi spendiamo in stipendi il 90 per cento: di tutte le risorse che il contribuente mette a disposizione del sistema universitario. Nel periodo 2001-2009 il Fondo di finanziamento ordinario è complessivamente cresciuto del 15,7

per il personale rispetto al Fondo di finanziamento ordinario: un parametro minimale di sostenibilità che il legislatore ha indicato fin dal lontano 1997. Ebbene, è successo esattamente il contrario: più il Fondo di finanziamento ordinario statale cresceva, più cresceva l'incidenza degli stipendi su di esso. Oggi ben 36 università hanno sforato quel tetto al lordo dei correttivi prorogati di anno in anno e e 7 università superano quel parametro anche tenendo conto degli stessi correttivi. In altre parole questo significa che non solo tutto il Fondo di finanziamento ordinario se ne va in stipendi, ma che anche una parte delle risorse proprie dell'ateneo frutto della contribuzione studentesca, dei fondi di ricerca, dei contratti esterni - viene requisita per far fronte a tali spese. Potrei aggiungere altre cifre, che però certamente conoscete: la proliferazione delle sedi e dei corsi; l'aumento del numero di insegnamenti e di contratti di docenza; il numero abnorme di corsi di dottorato di ricerca, che in Italia contano in media 5,6 studenti per ciascun ciclo triennale, il che vuol dire meno di due studenti per anno, e sparsi dovunque, anche in sedi dove non è onestamente concepibile poter offrire formazione a livello dottorale. Non posso però fare a meno di aggiungere almeno un altro dato. Nel suo primo Documento di programmazione economico-finanziaria l'allora ministro del tesoro Padoa-Schioppa ebbe a scrivere parole lungimiranti: il sistema universitario non poteva aspettarsi nuove risorse, ma doveva imparare a spendere meglio quelle che già riceveva: parole che condivido in pieno. Era la primavera del 2006, tempi di vacche grasse, non di recessione. Eppure, per il terzo anno della programmazione triennale, il 2008, il Governo di allora aveva previsto una riduzione del Fondo di finanziamento ordinario di 260 milioni.

Tanto preoccupato era il Tesoro su come sarebbero stati spesi quei denari da imporre la firma congiunta al decreto annuale di ripartizione. Non aveva torto. Oggi la maggior parte di quel Fondo - ben 468 milioni su 550, vale a dire l'85 per cento è assorbita dalla crescita stipendiale automatica del personale universitario, cosicché per le misure volte a rafforzare la qualità sono rimaste appena le briciole. Dietro tutti questi fenomeni si annidano due pericolose mistificazioni: l'illusione, o per meglio dire la presunzione, che per le istituzioni accademiche la sostenibilità economica non sia un requisito necessario e la strana idea che il numero dei docenti e la loro distribuzione geografica e disciplinare debbano essere parametrati sulle aspirazioni dei docenti stessi o di chi aspira a diventarlo, non sulle effettive esigenze e possibilità del sistema nazionale. Non è così, e non può e non deve essere così. L'università è un servizio pubblico largamente finanziato dal contribuente, e al contribuente deve rendere conto delle proprie scelte. Anzi, la solidità finanziaria è garanzia primaria di indipendenza: chi ha bisogno di prestiti, di piani di rientro, di contributi eccezionali, di salvataggi *in extremis*, rischia inevitabilmente di contrarre obbligazioni che minano il bene più prezioso per un ateneo: la sua autonomia. *(Applausi esplosione dei costi sarebbe in teoria anche accettabile - il che non vuol comunque dire sostenibile - se fosse stata accompagnata da un deciso e riconosciuto innalzamento della qualità media delle nostre università. Sono la prima a riconoscere, come dicevo, i meriti dei nostri atenei, che non sono pochi, ma sfido chiunque ad affermare che oggi le nostre università siano nettamente migliorate rispetto a dieci anni fa. Di fronte a questa situazione, onorevoli senatori, è necessaria un'assunzione di responsabilità collettiva: è quella che abbiamo oggi di fronte nel momento in cui dobbiamo esaminare e approvare questo disegno di legge. Il disegno di legge è indispensabile se vogliamo dare un contributo concreto ad un processo di risanamento di cui già si intravedevano i primi segni. Nei due anni che ci separano dalle linee guida, le nostre università non sono state ferme. Pur in un contesto non facile, hanno continuato a svolgere la loro insostituibile missione di insegnamento e di ricerca e soprattutto hanno avviato importanti azioni di riforma: hanno messo mano alla *governance*, accorpato i dipartimenti, eliminato corsi di laurea superflui, chiuso sedi decentrate insostenibili. Il Ministero, per parte sua, ha riunito molte scuole di specializzazione medica, al fine di raggiungere una massa critica soddisfacente, condizione essenziale di qualità. L'ANVUR (Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca) avrà dopo l'estate il suo primo consiglio direttivo. Il nuovo regolamento sui dottorati di ricerca

che segnala l'esigenza di attivare corsi solo in presenza di un numero adeguato di docenti e di chiudere i corsi con troppo pochi studenti. Tutte queste misure di razionalizzazione - mi preme ribadirlo - non servono solo per evitare sprechi ingiustificabili, ma prima di tutto per ragioni di serietà accademica. Tutte le patologie gestionali ed economiche ampiamente note e lamentate corrispondono infatti ad altrettanti cedimenti sul piano della qualità scientifica e didattica, che abbiamo il dovere inderogabile di garantire ai nostri studenti. Ma al di là di ogni misura tecnica e amministrativa, dobbiamo essere consapevoli che solo una vera riforma del nostro sistema universitario può consentirci di raggiungere nuovi traguardi. Il vero rischio che corriamo oggi è di far pagare gli errori del passato a chi non ne ha colpa: ai ricercatori e agli associati che non hanno sfruttato le promozioni facili degli anni scorsi e si trovano oggi di fronte a piramidi rovesciate difficili da scalare; ai dottorandi e agli assegnisti che vorrebbero portare nel sistema le loro competenze e il loro entusiasmo e trovano l'ingresso sbarrato; agli studenti, i più danneggiati dallo scadimento della qualità di alcuni corsi. Questo è un rischio che non intendo correre, come - ne sono convinta - non lo vuole nessuno di voi. Per evitarlo dobbiamo proporre soluzioni realistiche e serie, non illusioni. Pensare che il Fondo di finanziamento ordinario e l'organico possano crescere senza fine, come se fossero variabili indipendenti, è insieme una follia e un inganno, a cui dobbiamo reagire mettendo al centro del nuovo sistema la valutazione del merito dei singoli, in un quadro di doverosa sostenibilità economica, rispetto alla quale - ripeto - il Governo ha assunto un impegno. Onorevoli senatori, abbiamo di fronte a noi tempi non facili e sfide complesse, ma possiamo farcela se ci impegniamo in un nuovo «Patto nazionale per l'università», che propongo a questa Assemblea. Per i docenti dobbiamo creare un sistema che non proceda a fughe in avanti nel reclutamento seguite da lunghe carestie, ma sappia dosare le sue risorse in modo da garantire possibilità di accesso e di crescita regolari nel tempo, con cadenze certe e prevedibili. Per gli studenti dobbiamo insistere sulla necessità di offrire corsi di livello elevato nei contenuti e nelle modalità di erogazione, anche scoraggiando l'inseguimento di lauree magari facili, ma deboli sul piano scientifico e inutili per trovare un lavoro. Per il Paese, soprattutto, dobbiamo costruire un'università che goda pienamente della fiducia di tutti, cui sia riconosciuto fino in fondo il suo ruolo - unico ed insostituibile - di luogo primario della ricerca e di motore dello sviluppo sociale, economico e tecnologico. Per tutti questi motivi, mi auguro che sia ancora possibile un accordo tra maggioranza ed opposizione su alcuni punti qualificanti: penso alla presenza di prestigiosi esponenti della società civile nei consigli di amministrazione; al ruolo centrale affidato ai dipartimenti; alla revisione delle norme su tempo pieno e definito; alla centralità della valutazione per allocare le risorse; all'accorpamento dei settori scientifico-disciplinari; all'abilitazione scientifica nazionale a numero aperto; alla distinzione tra reclutamento e promozione, accompagnata nel transitorio da norme specifiche per agevolare la chiamata dei ricercatori di ruolo; alla limitazione nell'uso dei contratti di insegnamento per evitare che diventino fonte di precariato; alla struttura stessa dei nuovi ricercatori (*tenure track*). Sono tutti temi importanti ed ineludibili, se crediamo veramente nelle grandi potenzialità del sistema universitario. Restano alcune differenze ma, francamente, non tali e non tante da far comprendere un atteggiamento ostile al disegno di legge nel suo complesso. Né mi sento di condividere una posizione negativa sul disegno di legge motivata esclusivamente o principalmente dalla mancanza di fondi. È vero e l'ho detto: i fondi sono e restano un problema che dobbiamo risolvere, ma questo significa forse che dobbiamo rinunciare a qualunque idea di riforma? Siccome non ci sono garanzie sui fondi è meglio tenere bloccato, anche a livello normativo, il reclutamento, continuando ad essere l'unico Paese al mondo in cui non esiste un modo per diventare professori di università? È meglio tenerci le mille forme di precariato non regolato che affliggono i nostri giovani? Rinunciare a nuove regole chiare e trasparenti sulla valutazione? Di risorse aggiuntive ne abbiamo avute in quantità nello scorso decennio, grazie a Governi di centrodestra e di centrosinistra: è sotto gli occhi di tutti che il loro impatto non è stato positivo perché non è stato accompagnato dalle riforme necessarie. vi chiedo: se le riforme non si fanno né quando le risorse aumentano né quando le risorse diminuiscono, allora, onorevoli senatori, quando si possono fare? Esiste in questo Paese un tempo per le riforme? La mia risposta è: oggi. Oggi abbiamo di fronte a noi un'occasione irripetibile ed è nostro dovere coglierla fino in fondo, senza tentennamenti!

dal Senato, che si era concluso all'inizio del mese di maggio di questo anno. Ricordo brevemente le note più importanti del provvedimento in Esso contiene disposizioni di grande rilevanza in ordine all'assoluto divieto, per i neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente

a questo fine, per ottenere una patente professionale, occorre un attestato di non abuso di alcol e di non uso di sostanze di tipo stupefacente. Questa norma, che è molto chiara e netta, è stata fortemente condivisa sia dalla Camera che dal Senato. A fianco a questa forte disposizione, vi è anche però qualche segnale di apertura nei confronti dei giovani, come l'introduzione della guida accompagnata a 17 anni.

e poi devono essere accompagnati da persone con almeno dieci anni di patente. rilevanti che riguardano l'autotrasporto e che penalizzano ulteriormente i trasportatori che non rispettino il periodo

al lavoro di pubblica utilità in sostituzione di pene detentive e pecuniarie; ci sono norme che offrono la possibilità

previsione del riparto dei proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie. In particolare, la norma che riduce i proventi per gli enti locali, fatta peraltro in accordo con l'Associazione nazionale Comuni italiani, assegna una quota del 50 cento dei proventi delle multe per eccesso di velocità, comunque, allo Stato. Sotto questo profilo, la Camera, che ha in questo senso migliorato il testo licenziato dal Senato, ha ribadito la

in parte al Ministero delle infrastrutture, per gli interventi in ordine alla manutenzione degli impianti e delle infrastrutture, in parte al Ministero dell'interno, per il miglioramento dei controlli e della dotazione delle forze di polizia stradale,

Si è previsto, sempre a titolo di prevenzione, l'impiego di precursori nei locali che somministrano bevande alcoliche per dare la

in cui si ha l'uso o il possesso di un veicolo. C'è una norma di civiltà, peraltro mantenuta dalla Camera, che riguarda la possibilità di derogare al codice non soltanto

di essere soccorsi e trasferiti presso veterinari o strutture dedicate agli interventi di urgenza. Vi sono

La Commissione ha ritenuto tuttavia di non dover apportare ulteriori modifiche al testo, anche e soprattutto perché

come gli altri codici, un cantiere in continua evoluzione, anche per le evoluzioni tecnologiche che attengono sia agli impianti infrastrutturali che ai veicoli.

precisazioni che riguardano l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Qualora il provvedimento

l'entrata in vigore delle nuove norme, che riteniamo sicuramente utili per aumentare la sicurezza sulle nostre strade. Questa è la ragione

Signor Presidente, onorevoli senatori, credo che con questo provvedimento

legislatura, come ha detto il senatore Cicolani, con quattro passaggi in Parlamento, ma con una grandissima e bellissima disponibilità dei Gruppi,

La sicurezza stradale, com'è noto, ha tre componenti fondamentali. Innanzitutto che incidono sulla sicurezza stradale: noi purtroppo lamentiamo un *gap* nella costruzione di infrastrutture stradali che influisce sulla quantità di incidenti nel nostro Paese.

dell'incidentalità nel nostro Paese, compresa quindi la mortalità che è il punto più alto, assommi ad oltre 30 miliardi di euro. Se noi sommiamo a questi 30 miliardi di euro che costa al Paese in termini economici l'incidentalità, la perdita di vite umane, di un patrimonio di energie, di intelligenza e di forza, forza, il *gap* logistico del nostro Paese, che viene calcolato in altri 40 miliardi di euro l'anno, vediamo quanto sia importante il lavoro che si può portare avanti nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, e come questo debba essere uno delle priorità all'attenzione del Parlamento e della politica. Il senatore Cicolani ha già esaminato molto bene i contenuti più importanti del provvedimento. Ne segnalo alcuni per il mio incarico specifico, di cui sono particolarmente orgoglioso, e ringrazio il Parlamento per il lavoro che ha svolto sotto questo punto di vista. Abbiamo già detto che la norma che fa notizia è «chi beve non guida

per gli autisti professionisti al modello europeo: i nostri autisti, quando sono all'estero, se vengono fermati dalle forze dell'ordine, vengono sanzionati e se non pagano immediatamente,

All'interno di questo provvedimento, ci sono norme importantissime che sanzionano questi comportamenti, che hanno poi riflessi sulla sicurezza stradale. Un'altra norma è quella della targa personale; un'altra ancora,

però il fatto che questo provvedimento entri in vigore probabilmente già da questa settimana fa la differenza: sarà ben possibile dire

ma certo l'esito di quella discussione ha messo in evidenza che forse, tenendo in considerazione che la quarta lettura al Senato si sarebbe aperta a ridosso della pausa estiva, altro poteva essere il comportamento di assoluto buon senso che si sarebbe dovuto avere alla Camera. Sarebbe stata opportuna, per non dire indispensabile, una qualche forma di coordinamento maggiore tra le due Camere e in modo particolare tra le due Commissioni, per evitare che il combinato risultante dalla navetta parlamentare e dall'urgenza di far entrare in vigore il nuovo codice prima dell'estate finisse per demandare al Senato la sola funzione di ratifica di quanto già discusso, modificato e concordato altrove. È venuta a mancare in quest'occasione la capacità di elaborare un provvedimento comprensivo della visione più larga possibile. Proprio per questo eravamo inizialmente contrari all'assegnazione del testo in sede redigente, perché l'esame in Aula avrebbe permesso a tutti i parlamentari di trarre le proprie valutazioni sul merito del provvedimento. Certo, dalla mancanza di sicurezza sulla strada deriva per il nostro Paese una perdita insopportabile in termini di vite umane, di fronte alle quali forse passa in secondo piano la questione di come dovrebbero svolgersi i lavori parlamentari. Nel merito del provvedimento, tuttavia, è doveroso rilevare come le modifiche apportate alla Camera non siano marginali, nonostante - come si legge nei resoconti - fosse stato assicurato a tutti i deputati che tutte le ulteriori modifiche sarebbero state solo marginali e sempre votate all'unanimità. L'unanimità c'è stata per davvero; sulla marginalità delle modifiche si possono avere dubbi. Esse, in certi casi, vanno ben oltre il limite ed il merito della materia della sicurezza stradale. ad esempio, a quanto previsto all'articolo 54, che modifica la disciplina sulla somministrazione di alcool nelle ore notturne e, in particolare, prevede l'obbligo per gli esercenti di avere, presso ciascuna uscita del locale, un apparecchio di rilevamento del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcol. Così, intervenendo sul decreto-legge n. 117 del 2007, sono state riformulate le fattispecie vietate ed è stato ampliato e dettagliato l'ambito di applicazione della disciplina, prevedendo che debba essere interrotta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e che la stessa non possa essere ripresa nelle tre ore successive, salvo sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. la norma potrebbe anche essere condivisibile, ma il fatto è che successivamente viene disposto che i predetti divieti non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio e nella notte tra il 15 ed il 16 agosto. se la finalità della norma è quella di evitare che dalla vendita di alcolici prolungata nelle ore notturne possano derivare incidenti dovuti alla guida in stato di ebbrezza, derogare a tali divieti la notte di Capodanno e di Ferragosto equivale a dire: «Ma sì, a Capodanno e a Ferragosto potete anche mettervi alla guida ubriachi». Nello stesso articolo si sono poste prima norme estremamente restrittive, poi si è stabilita una deroga in alcuni giorni a tali restrizioni e da ultimo si è proceduto ad autorizzare i concessionari demaniali di spiagge ad organizzare feste con somministrazione di alcolici dalle ore 17 alle ore 20. Viene da chiedersi se la guida in stato di ebbrezza sia un pericolo solo nelle ore notturne. Non marginale mi sembra poi la soppressione della norma che prevedeva agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli per disabili e del tutto insensata appare la soppressione del divieto di superare i 60 chilometri quando su un motociclo si trasporta un minore, o ancora l'abolizione del casco obbligatorio in bicicletta per i bambini fino a 14 anni. È questa l'idea di prevenzione e di sicurezza che Nonostante le criticità ricordate, occorre riconoscere che sono stati apportati miglioramenti, come quelli relativi alle disposizioni sulla guida per i minorenni e alle relative sanzioni, così come al ripristino delle disposizioni sui programmi di educazione stradale nelle scuole e alla destinazione dei proventi delle multe. Ma il nostro voto parte dalla convinzione che la sicurezza non si può ottenere soltanto introducendo norme estremamente restrittive o inasprendo le sanzioni, che di per sé non sono in grado di costituire il sufficiente deterrente ai comportamenti di guida pericolosa. Pensiamo, in estrema sintesi, che i nodi sui quali occorre agire siano: il sistema di governo della sicurezza stradale; gli strumenti e le procedure per il coordinamento; il potenziamento dell'azione di controllo; la formazione e la cultura della sicurezza stradale; il monitoraggio degli interventi, dei risultati e delle sanzioni (articolo 208 del codice e il potenziamento del piano nazionale della sicurezza stradale. Di tutto questo c'è solo qualche traccia nel presente provvedimento. Da un lato, infatti, per sua stessa natura la sicurezza stradale è materia complessa che compete a tutti i livelli di governo e le cui scelte rimandano a questioni di fondo del sistema Paese, quali i trasporti e la mobilità, la rete infrastrutturale, il sistema produttivo. Essa necessita quindi di un approccio coerente, unitario, riconoscibile e riconosciuto nei diversi centri decisionali. Una riforma vera in materia di sicurezza stradale deve dare piena attuazione al principio di cui al comma 1 dell'articolo 2 del codice della strada, che pone come fini prioritari il perseguimento della sicurezza stradale, la riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare ed il miglioramento del livello della qualità della vita dei cittadini, eliminando o correggendo tutte le norme che siano in contrasto con il principio C'è bisogno di una riforma che favorisca la diffusione dei sistemi di mobilità alternativa e sostenibile, che possa garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada (l'Italia è un Paese dove ancora non c'è una cultura diffusa della sicurezza stradale) che orienti utenti, tecnici e decisori verso comportamenti responsabili ed efficaci. È decisivo, secondo noi, che il Paese faccia una scelta inequivocabile a favore della mobilità collettiva rispetto a quella individuale, del sistema dì trasporto pubblico rispetto a quello privato. Un'azione di questo spessore farebbe affrontare tutte le questioni a monte e a valle della sicurezza stradale con modalità decisamente inedite per questo Paese, anche se va detto che le recenti scelte, relative ad esempio - ma non solo - al trasporto ferroviario, non sembrano andare proprio in questa direzione. In altri termini, verrebbero affrontate in modo organico e coerente le problematiche a monte rete infrastrutturale urbana ed extraurbana, ai sistemi informativi e di controllo, dalla struttura dell'offerta di mezzi di trasporto alla domanda del loro utilizzo), come a valle (dall'organizzazione delle interconnessioni tra le varie scelte modali, all'educazione al loro uso, alla coerenza delle politiche assicurative, alla repressione della guida in stato di ubriachezza). Con una netta opzione per la mobilità collettiva, la vita umana sarebbe meglio tutelata, ma ne trarrebbe beneficio anche il sistema economico nel suo complesso, dato che con un progressivo decongestionamento sia delle grandi reti di collegamento sia della viabilità della città le relazioni umane ed economiche verrebbero facilitate e incentivate.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, innanzi tutto una premessa fondamentale: garantire la sicurezza sulle nostre strade è una necessità che appoggiamo e condividiamo pienamente. Ciò che non condividiamo è il cambiamento continuo della normativa, perché riteniamo che questo causi confusione e grossa incertezza tra i cittadini. Oltre a ciò, non condividiamo il continuo inasprimento delle sanzioni, perché ciò non garantisce maggior sicurezza e non è socialmente difendibile, perché mette in seria difficoltà economica cittadini che hanno già difficoltà ad arrivare a fine mese. Diversamente dalle altre Regioni italiane, in Trentino-Alto Adige/Südtirol i sono molti e rigorosi e le norme e le sanzioni vengono applicate alla lettera. Anziché inasprire anno dopo anno le sanzioni, consiglierei dei controlli mirati su tutto il territorio nazionale.

dalle tre di notte in poi, evitando così vendite incontrollate fuori dai locali notturni. Mi rincresce, invece, che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati siano state cambiate alcune norme introdotte da noi in seconda lettura e per le quali ci eravamo battuti. Un esempio tra tanti è l'articolo riguardante la restituzione della patente D. In Senato, grazie anche all'apporto

alla Camera tale limite è stato invece abbassato a 68 anni e sono stati previsti ulteriori obblighi burocratici per la restituzione della patente. Potrei fare altri esempi, ma mi limito a ribadire che la sicurezza sulla strada si garantisce con l'educazione stradale, con campagne di sensibilizzazione: in una parola, con la prevenzione.

modifiche sui ciclomotori e sulle minicar. Questo è già stato sottolineato da chi mi ha preceduto: si tratta sicuramente di un intervento migliorativo, e non c'è bisogno che mi addentri nelle motivazioni che mi fanno considerare

solo che nello stesso momento in cui andiamo a dire a tutti che bisogna andare in pensione più tardi perché le aspettative di vita si sono allungate, andiamo invece a dire a qualcuno (che magari utilizza ancora la patente

non possono essere utilizzati o installati fuori dai centri abitati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità. Questo, personalmente e a nome del mio Gruppo, ritengo che sia sicuramente un intervento migliorativo.

la Camera ha soppresso la disposizione che consentiva alle biciclette la sosta sui marciapiedi all'interno delle aree pedonali in mancanza di strutture idonee di parcheggio. Si potrebbe discutere ancora per ore e per giorni su questa disposizione, dell'introduzione dell'obbligo di seggiolini per il trasporto sui veicoli a due ruote di minori di 12 anni

Anche questa è una norma che avevamo introdotto al Senato dopo ampi ragionamenti riguardo alla volontà di assicurare una protezione a chi usa un mezzo (che potrebbe sembrare innocuo o banale) come la bicicletta. Nel momento stesso in cui avviene una caduta

corretta relativa all'aumento di un terzo delle sanzioni pecuniarie per le violazioni commesse tra le ore 22 e le ore 7, e quindi nell'orario notturno, per i casi di guida con tasso alcolemico compreso tra lo 0,5 e lo 0,8 Ritenevamo fosse una norma importante, perché comunque condizionava pesantemente chi guida in stato di ebbrezza in quegli orari.

Grazie,

non sono mai venute meno, in ragione dell'interesse generale per la materia trattata, ossia la riduzione dell'incidentalità stradale, con la conseguente salvaguardia ed incolumità di vite umane. senso di responsabilità è dovuto anche per un fattore tempo, che ha alimentato una legittima attesa nelle migliaia di operatori della strada, di fronte a un'incertezza normativa che chiedeva di essere risolta, anche per rispetto dei milioni di utenti della strada, alla vigilia del solito esodo massivo sulle nostre strade. Il tempo di approvazione di un provvedimento in generale, e di questo in particolare (com'è stato ricordato anche dal Sottosegretario), non è mai, infatti, un fattore secondario per la valutazione di qualità del provvedimento stesso. Un provvedimento, quello in questione, giunto ormai alla sua quarta lettura, dopo oltre 20 mesi di gestazione solo in questa legislatura e oltre un anno, maturato senza successo, in quella precedente. Molte delle norme - che sono state richiamate - presenti nel provvedimento possono infatti essere giustamente ritenute un lascito della precedente legislatura, a richiamo del fatto che da tempo sulla materia prevale un corretto atteggiamento *bipartisan*, che sostanzialmente ci sentiamo di confermare anche in questa legislatura, pur partendo da approcci culturali sensibilmente diversi e perseguendo obiettivi talvolta non simili. Desidero infatti confermare in questa circostanza un sincero apprezzamento per la sensibilità e l'attenzione dimostrata dal relatore e dal Governo; in particolar modo un ringraziamento va alla generosa disponibilità dimostrata dalla struttura ministeriale, e ovviamente dal Presidente; un aspetto, questo, non formale né rituale, credo sia di grande valore per la politica e le istituzioni del nostro Paese, specialmente in un periodo di grande turbolenza come quello che stiamo attraversando. Ciononostante, non possiamo non sottolineare, proprio in ragione del richiamato senso di responsabilità e della più volte enunciata comunione d'intenti, che il provvedimento contiene elementi per noi non condivisibili nell'approccio e nel metodo perseguito, ma anche purtroppo nel merito di alcune norme contenute nel testo in approvazione, che hanno a nostro avviso determinato un sensibile scarto

dell'intero codice della strada: riscrittura che probabilmente da oggi si rende ancora più urgente, perché la stratificazione della produzione normativa registrata dal 1992 ad oggi ha finito per rendere ormai incomprensibile quello che forse è il codice di maggior uso e consumo da parte dei cittadini, ma anche perché occorre davvero renderlo più flessibile nel recepimento delle sempre più frequenti e necessarie direttive comunitarie, senza per questo modificarne ogni volta l'impianto principale, ma conferendo alle norme secondarie e regolamentari i principali aspetti dispositivi; in ultimo, perché meglio sarebbe stato se il legislatore si fosse concentrato in un'opera di indirizzo per il nuovo codice che potesse essere propedeutica anche ai futuri obiettivi comunitari in termini di sicurezza stradale. stesso modo, forse sarebbe stato più saggio se il Governo, forte delle due letture parlamentari, avesse anticipato con un proprio decreto il corpo delle norme approvate di fatto da entrambe le Camere, per consentire la correzione di alcuni aspetti che invece il Senato - come è stato ricordato - è stato costretto forzatamente e ingiustamente a digerire, ma anche per consentire un primo impianto di norme riguardanti l'autotrasporto,

abbiamo espresso: in quella circostanza è stata veramente persa un'occasione. Con tutto ciò, non abbiamo difficoltà a riconoscere che sussistono aspetti contenuti nel provvedimento approvato in terza lettura alla Camera che lo migliorano sensibilmente, in particolare su un punto per noi non secondario, come la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative. Secondo una logica assolutamente condivisibile, le risorse provenienti dalle infrazioni al codice della strada devono prioritariamente essere finalizzate all'innalzamento della sicurezza stradale, e ciò non come principio normativo fino ad oggi sistematicamente disatteso o eluso, ma come norma e procedura cogente e vincolante. conclusione, non possiamo però far velo agli elementi a nostro avviso distonici che non ci consentono di avere un giudizio complessivo condiviso sull'intero provvedimento. Si tratta di norme che, proprio in ragione della terza lettura della Camera, come è stato ampiamente ricordato da chi mi ha preceduto, disapplicano disposizioni di buon senso introdotte proprio dal Senato e che purtroppo abbassano pericolosamente il livello di sicurezza stradale. Mi riferisco alla cancellazione del limite massimo di velocità di 60 chilometri orari per motociclisti che trasportano minori, o alla cancellazione della norma che per i minori fino a 14 anni avrebbe imposto l'uso del casco anche sulle biciclette. una norma importante, anche per l'indubbio valore simbolico ed educativo per le nuove generazioni in termini di sicurezza stradale, a partire proprio dall'uso delle dotazioni strumentali di prevenzione per la sicurezza e l'incolumità personali. Disappunto e dispiacere esprimiamo anche per il ripristino a 90 e 100 giorni del termine consentito per la notifica del verbale di accertamento dell'infrazione: ciò è assolutamente incomprensibile ed inconcepibile, in una società telematica come la nostra. In ultimo, ma non certo per importanza, critichiamo le modifiche al provvedimento che hanno recepito l'iniziale cosiddetto emendamento Giovanardi, teso a disciplinare esercizi commerciali, ma non solo, anche stabilimenti balneari, ma non solo, e perfino i circoli (e magari anche le parrocchie!) che a vario titolo vendono e somministrano bevande alcoliche e superalcoliche. Colleghi, sia chiaro: siamo consapevoli che il legislatore - cioè tutti noi - va a fissare con questo provvedimento solo limiti probabilmente provvisori, e sicuramente parziali, alle condizioni di guida in stato di ebbrezza, e che probabilmente in futuro ci potrà essere anche maggiore intransigenza, nei registri di una prossima riforma, all'insegna del principio come è stato ricordato - per cui chi beve non guida. Tuttavia, altra cosa è prevedere norme dall'anacronistico sapore proibizionistico che -non per principio ideologico, ma perché l'esperienza ne ha sempre decretato un esito fallimentare - sono fuori dalla storia e dalla cultura del nostro Paese e che, quando sono state introdotte, non hanno tardato a sortire effetti opposti a quelli attesi.

affida invece alla prevenzione, all'educazione, all'informazione, ma soprattutto ai controlli stradali, che ci vedono ancora troppo lontani rispetto alla media europea dei Paesi più virtuosi in termini di sicurezza stradale. Di controlli stradali e del loro incremento, in questo provvedimento, purtroppo, non vi è traccia, come avremmo invece voluto. Per tutti questi motivi, il Gruppo del Partito Democratico è costretto, davvero con dispiacere, a distinguere il proprio voto conclusivo con un'astensione.

Come hanno ricordato quasi tutti i colleghi che mi hanno preceduto, arriviamo a questa conclusione portando a compimento due risultati, ai quali anch'io attribuisco molta importanza. Il primo risultato

della strada, dopo che per molto tempo, anno per anno, si è cercato di emendarlo con interventi settoriali, categoriali e marginali. Oggi, invece, siamo alla conclusione di un lungo *iter*,

Il secondo risultato, che anch'io sottolineo con evidente soddisfazione, è che tutto questo lavoro lo abbiamo fatto in una logica *bipartisan*. Il Governo è stato un utilissimo supporto, con i suoi uffici ed il ruolo del Sottosegretario, che ringrazio, e del Ministro, che pure ha seguito con grande attenzione questo *iter* in Commissione. attenzione questo *iter* in Commissione. Sono prevalse logiche per cui abbiamo cercato di evidenziare il ruolo propositivo del Parlamento, senza pregiudizi, con atteggiamento aperto, finalizzato a individuare le norme più efficienti e funzionali a raggiungere l'obiettivo che ci eravamo posti, cioè quello di

che in una condizione diversa non solo le proposte, ma anche le questioni emendative da lui poste in Commissione nel tentativo di correggere modifiche apportate dalla Camera, che anche a noi non sembrano, e non sono assolutamente da considerare, migliorative del testo, ci avrebbero visti assai più attenti e disponibili, se non fosse prevalso, anche per noi, il senso di responsabilità coniugato con i tempi stretti che abbiamo di fronte.

sulle questioni che interessano a milioni di cittadini, nonostante la confusione che appare sulle prime pagine di tutti giornali, il Parlamento ha ancora la capacità di individuare un punto di mediazione avanzato e quindi di privilegiare gli interessi generali del Paese a quelli di categoria e settoriali. Questo mi pare un risultato molto positivo all'interno di una legislatura che, non ce lo nascondiamo, è purtroppo caratterizzata da tanti elementi di divisione e tentativi di forzatura, che sicuramente non qualificano l'attività del Parlamento. Grazie, che tutti attendono e che era bene diventasse legge, come ha ricordato il relatore Cicolani, prima dell'esodo estivo. Questo provvedimento, signor Presidente, è ancor più importante se lo mettiamo in relazione con una strategia che, mi permetto di dire

convenienti questi investimenti. Tuttavia, tutto sarebbe una risposta parziale se non lo coniugassimo con la necessità di rilanciare il sistema viario italiano, il sistema infrastrutturale e le autostrade del nostro Paese. Infatti,

necessitavano di una risposta diversa e probabilmente con il tempo ci sarà modo di correggere ancora il testo in tal senso. Oggi concludiamo questo *iter* approvativo, sapendo che il Parlamento esce a testa alta, perché fornisce all'opinione pubblica, a milioni di cittadini, al Paese intero delle certezze che si cercavano da anni

hanno dimostrato una sensibilità non comune nel privilegiare un confronto aperto su temi concreti, al rappresentante del Governo, sottosegretario Giachino, e confermo il voto favorevole del Gruppo del PdL. nuova finestra"). Come precedentemente comunicato, il voto finale del disegno di legge è rinviato alla giornata di domani, nell'orario che sarà tempestivamente comunicato ai Gruppi parlamentari.

su eventuale autorizzazione rilasciata dal Governo italiano, sia, con maggiore pericolosità, su autorizzazioni rilasciate da Governi degli Stati rivieraschi. rivieraschi. Il Mediterraneo è un mare ad altissima sensibilità di inquinamento da catrame pelagico, ma soprattutto è un mare talmente interno alle sue alle sue terre che qualsiasi eventuale danno si provocasse in qualsiasi punto dello stesso avrebbe effetti devastanti sull'intero sistema ambientale e sulle coste di tutti gli Stati rivieraschi.

ho chiesto di intervenire per manifestare la profonda preoccupazione per le vicende che riguardano la FIAT e, soprattutto, i suoi lavoratori e per il futuro di un'azienda che, nel nostro territorio, ha rappresentato l'industria in Italia. È paradossale che nelle prossime ore, all'incontro organizzato dal ministro Sacconi, non ci sarà il Ministro dello sviluppo economico. Mentre il PdL pensa a risolvere i problemi interni, il Paese va a rotoli. Siamo in piena crisi e la FIAT, per bocca dell'amministratore delegato Marchionne, trasferisce in Serbia la costruzione della nuova monovolume.

invece l'azienda torinese comunicherà la disdetta del contratto nazionale dei metalmeccanici. La verità è che questi signori non hanno il coraggio di dire di dire che hanno abbandonato ogni tipo di politica industriale. Alle centinaia di vertenza su migliaia di posti di lavoro - ce ne sono 200 che giacciono negli uffici del Ministero dello sviluppo rispondete decapitando le intercettazioni e impoverendo il Paese con una manovra che tutela i super ricchi. Volete chiudere i problemi di Termini Imerese, di Pomigliano d'Arco e di Mirafiori con il vostro assordante silenzio devastando i fondi per le aree sottoutilizzate e saccheggiando i fondi del Ministero delegato a inaugurare sagge politiche industriali. Venga il sostituto di Scajola in Aula, venga il Presidente del Consiglio qui, ci dica cosa fa il suo Governo per salvare questo Paese, ma non ci racconti bugie, farse e quant'altro. Ci spieghi perché sta smantellando la politica industriale del Sud e sta impoverendo il Paese. *(Applausi